l'estratto del mio intervento per fare una segnalazione alla procura della Repubblica di Roma, perché credo non sia più tollerabile che società di questo tipo intervengano sul dibattito del nostro Paese.

Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi discutiamo, recante nuove disposizioni in materia di aree protette nel

Il testo in questione, che tiene conto delle normative in materia di ambiente e in particolare della direttiva europea

nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione. Il testo in esame evidenzia la necessità di raggiungere degli obiettivi strategici previsti in sede ONU dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la conservazione del mare e delle risorse marine, l'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, adottando azioni efficaci e immediate per ridurre in modo determinante il degrado degli ambienti naturali,

La legge-quadro n. 394 del 1991 ha contribuito, anche grazie al lavoro svolto dalle istituzioni e dalle associazioni ambientaliste, a inquadrare in un contesto normativo i parchi e le aree protette. Queste ultime rappresentano una realtà molto estesa della nostra penisola: infatti, dai dati del 2010 riportati dalla banca dati delle aree protette, la superficie protetta

di superficie protetta a mare e circa 2.300 siti di importanza comunitaria (SIC), divisi in zone speciali di conservazione e in zone di protezione speciale Parliamo complessivamente di circa 24 parchi nazionali, 29 aree marine protette e 52 parchi regionali. anni dall'approvazione della legge quadro del 1991 e il contesto è profondamente cambiato. E se a livello istituzionale dobbiamo rispondere alle indicazioni europee che ci giungono dalla guida delle normative comunitarie, a livello ambientale sono cresciute l'attenzione e la presa di coscienza in tema di cambiamenti climatici e di tutela ambientale. Oggi siamo dunque davanti a una sfida globale che ci fa sentire ancora più determinanti nel voler intervenire nella lotta l'educazione alla sostenibilità e la valorizzazione dei territori e delle economie locali. Proprio quando parlo di inversione di marcia, intendo porre l'accento sulla necessità di modificare l'approccio con cui si accosta questo argomento: un argomento che dovrebbe interessare tutti i Comuni del nostro Paese e che rappresenta parte del nostro sistema economico. La gestione dei parchi e delle aree protette è uno strumento economico e sociale utile per l'intera comunità e può essere fonte di sviluppo e di integrazione per un territorio, ma solo e soltanto se si punterà a uno sviluppo ecosostenibile e verde. La salute del pianeta e dei nostri figli e le modifiche apportate al provvedimento che oggi discutiamo mirano a creare e a rafforzare le condizioni per migliorare gli aspetti funzionali e gestionali dei parchi italiani, promuovendo le buone pratiche e l'uso delle risorse naturali. Le aree protette devono rappresentare un patrimonio culturale comune e da parte nostra - mi riferisco all'intenso lavoro svolto in Commissione - tutte le parti politiche hanno voluto apportare un proprio contributo volto a migliorare l'anima del provvedimento. I parchi sono importanti nei nostri territori dove nascono; ormai sono diventati parte integrante di un'economia locale:

Entrando nel contesto del disegno di legge, abbiamo voluto snellire e semplificare la *governance* delle aree protette, eliminando le lungaggini che si verificano a causa dei commissariamenti e della farraginosità della burocrazia. Appare fondamentale rafforzare i poteri del presidente e tale rafforzamento dei poteri non permetterà la compatibilità con qualsiasi altro incarico elettivo o con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici. Con l'abrogazione dell'albo dei direttori di parco si avrà una procedura meno opaca e più immediata anche per la nomina del direttore, che sarà designato dal consiglio direttivo sulla base di una selezione pubblica tra profili di comprovata esperienza nella gestione delle aree protette. Anche la composizione del consiglio direttivo cambia: si passa, infatti, dagli otto ai dieci membri, che saranno designati per il 50 per cento dalla comunità del parco. Tutto questo serve per snellire, semplificare e rendere le decisioni più rapide e farà capo - come abbiamo sottolineato - alla figura del presidente nominato, il quale agirà in stretto contatto con la comunità del parco sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del La meta che vorremmo raggiungere è quella di avvicinare il parco al territorio e alla comunità, perché solo creando una comunicazione, un interscambio fra il territorio e gli abitanti si avrà una migliore conservazione dell'area protetta, degli *habitat* e delle biodiversità. Positiva è anche la proposta di istituire un nuovo comitato per le aree protette che metta assieme tutti i parchi nazionali e regionali, e che al suo interno veda il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quello delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, i Comuni, Federparchi e le associazioni ambientaliste, con l'egida e il supporto tecnico dell'ISPRA. L'ISPRA sarà dunque chiamato al supporto tecnico-scientifico, al monitoraggio, al controllo ambientale, e dovrà occuparsi di individuare gli strumenti operativi e valutare le modalità di intervento di qualunque genere nelle aree protette. Tale concetto - come si è detto - è stato ampliato nelle zone a protezione speciale, ai siti di importanza comunitaria e alle zone speciali di conservazione. signor Presidente, un ringraziamento va al relatore Caleo, per il lavoro che ha svolto e per la grande collaborazione che ha dato a tutti noi della Commissione ambiente, lavoro che ha permesso di dare seguito e voce alle richieste delle istituzioni locali, istituendo una nuova area marina protetta lungo lo specchio acqueo marino marino prospiciente all'area del parco naturale della terra di costa Otranto-Leuca, un piccolo ulteriore tassello per garantire la tutela del mare e dell'ambiente lungo uno dei tratti più belli della costa italiana. Con la speranza che al nostro segnale di apertura segua un altrettanto segnale da parte del Governo di apportare in futuro miglioramenti e modifiche al contesto normativo in materia di aree marine protette, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti annuncio il nostro voto favorevole sul provvedimento.

attraverso la tutela delle aree protette e degli ecosistemi, anche per la stessa conservazione della specie umana. Il nostro Paese detiene il primato europeo nella biodiversità ha una dotazione importante di *habitat*, molti dei quali dichiarati prioritari a livello comunitario. Tra parchi nazionali e regionali, aree marine protette e aree protette a livello comunitario risulta difeso quasi il 22 per cento dell'intero territorio nazionale. Si tratta di una ricchezza che occorre valorizzare adeguatamente, quale risorsa vera e propria del nostro territorio; un'opportunità di sviluppo, anche ai fini turistici e per la preservazione delle tradizioni e delle identità; si può trattare come un mero vincolo territoriale, tale da rappresentare un problema soprattutto alle attività economiche ubicate all'interno. Secondo il nostro Gruppo, le Regioni e gli enti locali, ossia le istituzioni più vicine alle necessità del territorio e dei cittadini, devono assumere un ruolo chiave, devono essere i soggetti responsabili della *governance* delle aree protette e della pianificazione paesaggistica. Qui invece si va nella direzione contraria. Una delle modifiche importanti proposte dal disegno di legge è la semplificazione per l'istituzione delle aree protette marine, prevedendo l'estensione dei parchi nazionali terrestri anche nelle aree protette marine contigue. Purtroppo, però, non si prevede la possibilità di istituire aree marine protette e riserve marine anche da parte delle Regioni, al fine di evitare per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali una doppia gestione con oneri a gravare con oneri a gravare sulle finanze pubbliche. Un altro concetto non condivisibile è l'individuazione di un territorio contiguo all'area del parco, che viene sottoposto alla *governance* dell'ente parco stesso. Non ci piace che il regolamento del parco possa disciplinare nelle aree contigue le attività della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, sottraendo competenze al Comune e alla Regione. anche se è comprensibile l'obiettivo di trovare finanziamenti per i bilanci dei parchi, vista la penuria delle risorse statali, non condividiamo l'imposizione delle *royalty* alle concessioni delle attività economiche presenti nelle aree protette e, addirittura, in quelle nelle aree contigue, che dovranno pagare, chiaramente correndo il rischio di essere messe in difficoltà economica. E che dire della tanto sbandierata dal Governo semplificazione dei procedimenti amministrativi? Da una parte si semplificano le disposizioni della conferenza di servizi; dall'altra parte, invece, si elimina il silenzio assenso sull'inerzia dell'Ente parco nell'esprimere il parere sugli interventi infrastrutturali, anche per i casi di interventi edilizi minori. Riteniamo che l'inerzia colpevole dell'Ente parco non debba e non dovrebbe determinare la paralisi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione. Un'altra questione che denunciamo è l'eliminazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle aree contigue del parco. Non si comprende la *ratio* della norma, dal momento che il disegno di legge estende appunto la *governance* e il regolamento del parco anche alle aree contigue, ma restringe la possibilità degli indennizzi nell'area del parco, eliminando peraltro i risarcimenti che potrebbero risultare più onerosi per gli enti parco, ma meno accettabili per i cittadini danneggiati. Il disegno di legge presenta anche disposizioni positive - non lo neghiamo - come la diminuzione degli organi degli enti attraverso l'eliminazione della giunta, la diminuzione dei membri del consiglio direttivo e dei revisori, e altro ancora. Ma, sempre in tema di *governance*, non si condivide il previsto silenzio-assenso sull'intesa con la Regione per la nomina del presidente dell'Ente parco. L'assenza dell'intesa della Regione per la nomina del presidente è in generale una centralizzazione della gestione in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela come anche la 1a Commissione, censurandola, ha definito «incongrua» questa disposizione. Con riferimento all'attività venatoria, la modifica è altamente penalizzante e umiliante per tutti i cittadini e cacciatori italiani, tra l'altro senza alcun bisogno, senza alcuna necessità, poiché ad oggi si è raggiunto un buon equilibrio fra aree protette e aree di caccia programmata. Sono inaccettabili le modifiche che danno in pratica la gestione completa dei siti Natura 2000 agli enti gestori dei parchi, anche se esterni all'area protetta, e li trasforma tutti in aree contigue ai parchi e alle riserve. Mentre a legge vigente la caccia nelle aree contigue alle protette viene disciplinata dalle Regioni, con l'articolo 5 si stabilisce invece che la regolamentazione spetta all'Ente parco, e addirittura con il parere dell'ISPRA che, nel caso delle aree protette regionali, diventa vincolante. Mentre a legge vigente il parco, accertati squilibri ecologici, può tentare di ricomporli con prelievi faunistici e abbattimenti selettivi, autorizzando in pratica la caccia, con la modifica viene inserito esplicitamente il divieto assoluto dell'attività venatoria nei parchi nazionali e regionali, rendendo pertanto chiara la volontà di proibire anche una eventuale deroga mediante il regolamento del parco. È chiaro a tutti che la modifica è stata fortemente voluta e sponsorizzata da tutte le associazioni ambientaliste e animaliste di sinistra, che porterà a un accentramento assoluto del potere nelle mani del Ministero dell'ambiente e della tutela con il conseguente completo svilimento di qualsiasi potere decisionale e gestionale degli enti locali presenti sul territorio ove i parchi ricadono. Questo non ci piace. Non solo è contro la tutela delle tradizioni culturali e identitarie dei nostri popoli che vivono in questi luoghi che oggi si chiamano parchi, ma è anche contro ogni logica di federalismo e decentramento. Colleghi, guardate che la centralista riforma costituzionale ha avuto il via libera solo nei vostri sogni, perché dalla sera del 4 dicembre dovrete fare i conti con una realtà ben diversa da quella da voi auspicata. Sull'istituzione del Parco del Delta del Po, con tanto di relativa delega al Governo, ribadisco in sintesi la posizione del Gruppo della Lega Nord già espressa ampiamente ieri, in occasione della dichiarazione di voto di astensione all'articolo 25, che rispecchia la volontà delle istituzioni e delle comunità del territorio locale. C'è la contrarietà assoluta all'ipotesi di parco nazionale: la *governance* deve rimanere in capo ai territori. Non è accettabile che il costituendo parco unico sia prodromico alla nascita di un parco nazionale, come ha affermato il relatore Caleo, nonostante il collega Vaccari abbia cercato di sminuire. Vi è contrarietà netta all'ampliamento della superficie del parco e all'introduzione di nuovi vincoli sul territorio. Il parco deve essere interpretato non come camicia di forza, ma come elemento di sviluppo e promozione del territorio e delle attività umane in esso esistenti, in particolare la pesca, la vallicoltura, l'agricoltura e la caccia. Dovrà, infine, esserci il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali e delle categorie produttive. Non verrebbe mai accettato un parco frutto della sola visione delle associazioni ambientaliste e che scavalchi i rappresentanti istituzionali ed economici del territorio. Mi avvio alle conclusioni, Presidente. Avevo detto in discussione generale che il Gruppo Lega Nord-Autonomie si sarebbe posto in attenta osservazione della fase emendativa per le valutazioni e le considerazioni finali sul provvedimento. Purtroppo, tutti i nostri emendamenti sono stati respinti, lasciando permanere nel testo, oltre alle luci (poche), molte ombre, che portano persino a peggiore la legge quadro delle aree protette. Le Regioni e le Province autonome vengono sempre più private di potere, persino con disposizioni che limitano le prerogative costituzionalmente riconosciute loro in materia, come ha sottolineato e anche denunciato la 1a Commissione permanente. Si tratta, dunque, di una ulteriore centralizzazione che va nella direzione opposta a quella auspicata e tracciata in passato, nella precedente legislatura, dalla Lega Nord. che, purtroppo, il nostro Gruppo, prendendo anche atto del lavoro fatto in questa Assemblea, voterà contro al provvedimento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da più parti abbiamo sentito affermare in quest'Assemblea che le aree protette nel nostro Paese rappresentino uno scrigno di bellezza, valori paesaggistici, biodiversità ricchissima, ma anche di cultura, tradizioni agroalimentari, storia. E questo risponde certamente a verità. Ecco perché possiamo con tranquillità affermare che, a partire dalla legge quadro n. 394 del 1991, la storia della tutela del patrimonio naturale italiano aveva tutte le premesse per essere positiva. A questa legge va, infatti, il merito di aver messo in piedi - per la prima volta - un vero

ed è progressivamente mutato l'atteggiamento delle popolazioni riguardo ai territori protetti. Quindi, la situazione è certamente migliorata rispetto agli anni Novanta. Infatti, l'Italia è il Paese europeo che ha istituito il maggior numero di aree protette in Europa. Ciò è servito in parte a limitare la cementificazione e il consumo di suolo. Dobbiamo però dire che le potenzialità della legge n. 394 non si sono potute esprimere compiutamente, per diverse ragioni come - per esempio - l'atteggiamento della politica, che ha cercato negli anni di snaturare in qualsiasi modo il ruolo che con che con chiarezza invece la legge aveva attribuito a parchi e riserve, e cioè di perseguire una missione di conservazione e promozione dei valori naturalistici. L'altra ragione è legata alle risorse economiche, che sono diventate sempre più scarse, mettendo i parchi sempre più in difficoltà rispetto alle funzioni da assolvere, situazione che si è amplificata con l'adesione agli ultimi trattati europei. Pertanto, una riforma sulla gestione di parchi e aree protette era sicuramente opportuna, alla luce del tempo trascorso, ma una riforma che puntasse alla rimozione delle criticità emerse in venticinque anni: dalla politicizzazione degli enti gestori ai problemi finanziari, strutturali e gestionali delle aree protette; per non parlare della necessità di fare un punto sul coinvolgimento delle popolazioni locali. A questo fine la domanda che occorre porsi è la seguente: i ritardi e le mancanze che abbiamo registrato in questi anni sono dovuti veramente a difetti normativi oppure sono addebitabili più che altro a ragioni politiche? Solo partendo da una risposta concreta possiamo sperare che le aree protette possano diventare parte di un processo

se non ci sarà uno sforzo autentico per rendere efficaci queste norme sul terreno dell'applicazione concreta, potremmo trovarci di fronte all'ennesima delusione a riprova del fatto che qualunque buona legge, se non trova terreno fecondo nella sua operatività quotidiana, può risultare improduttiva degli effetti sperati, se non addirittura dannosa. Pertanto, a nome del gruppo Grandi Autonomie e Libertà, e nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo, annuncio il mio voto di astensione. Presidente, onorevoli colleghi, dall'approfondito dibattito cui abbiamo partecipato in quest'Aula un dato emerge pacifico, la *mission* delle aree protette è costituire strumenti per la tutela della biodiversità, del paesaggio, delle formazioni geologiche e dei beni comuni in esse situati, nonché strumenti per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo territorio deve essere posto in relazione con la matrice territoriale di area vasta attraverso le reti ecologiche e la pianificazione paesaggistica, perché la valorizzazione del patrimonio naturale riguarda non solo la valorizzazione economica, ma anche il riconoscimento del valore materiale e immateriale del patrimonio naturale e paesaggistico, dell'ecosistema e dei beni La strategia dell'Unione europea sulla biodiversità prevede di arrestare la perdita di biodiversità entro l'anno 2020. In questo senso la revisione della legge n. 394 del 1991, anche con la volontà manifesta di creare nuove aree protette, costituisce un indicatore sensibile per comprendere per comprendere se il nostro Paese sia sulla buona strada per dare una mano al raggiungimento degli obiettivi europei. Certamente sono stati compiuti molti progressi in tanti settori, ma si evidenzia la necessità di sforzi più intensi per tener fede agli impegni assunti dagli Stati membri La capacità della natura di pulire l'aria e l'acqua, impollinare le colture e limitare l'impatto di catastrofi quali le inondazioni, è compromessa, con potenziali costi elevati e imprevisti per la società e per la nostra economia. Un sondaggio d'opinione a livello europeo, pubblicato di recente, conferma che la maggioranza dei cittadini europei è preoccupata per le conseguenze della perdita di biodiversità ed è consapevole delle ripercussioni negative che questo fenomeno può avere sulla salute e il benessere della specie umana e, quindi, anche sul nostro sviluppo economico a lungo termine. In primo luogo, gli Stati membri devono attuare meglio la legislazione europea in materia di protezione della natura. Più dei tre quarti dei principali *habitat* naturali nell'UE sono attualmente in condizioni insoddisfacenti, e molte specie sono a rischio di estinzione. arresto della perdita di biodiversità dipende anche da quanto efficacemente le questioni legate ad essa sono integrate nelle politiche interne in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca, sviluppo regionale e commercio. La riforma della politica agricola comune offre la possibilità di una maggiore integrazione delle questioni connesse alla biodiversità, ma la misura in cui gli Stati membri attueranno i provvedimenti a livello nazionale sarà decisiva per garantirne il successo. Infine, occorre riconoscere e apprezzare per il suo giusto valore il nostro capitale naturale, non solo entro i limiti delle aree protette ma in generale nel nostro territorio e nei nostri mari. Il ripristino degli *habitat* naturali e la costruzione di infrastrutture verdi continuano a rappresentare delle sfide per il nostro Paese. Questa strategia dovrebbe comportare vari benefici per una serie di settori, compresa l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Le specie esotiche invasive sono una delle minacce alla biodiversità che registra la crescita più rapida in Europa, causando danni significativi all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, con un costo nell'Unione europea pari ad almeno dodici miliardi di euro l'anno. Su scala mondiale, l'Unione europea contribuisce in ampia misura ad arrestare la perdita di biodiversità. Insieme ai suoi Stati membri, l'Unione europea è il principale donatore finanziario per la conservazione della biodiversità, ma è anche vero

e le aree protette, con la previsione che la gestione di SIC e ZPS possa essere affidata agli enti parco territorialmente vicini. Questo è un aspetto da non sottovalutare, perché i parchi sono gli unici soggetti che dispongono del *know how* e del personale specializzato necessario per la gestione di queste aree. Lo abbiamo detto in discussione generale e lo ribadiamo in questa sede: non possiamo che essere d'accordo con le norme di semplificazione e riduzione dei costi sugli organismi di gestione dei parchi. Siamo d'accordo con la soppressione della giunta del parco, come pure apprezziamo la norma che prevede l'incompatibilità per il presidente del parco con altre cariche istituzionali. D'altronde, ricoprire la carica di presidente del parco richiede un impegno talmente intenso da risultare poco compatibile con altre attività istituzionali. In quanto ai famigerati piani parco, poi, crediamo che costituisca una svolta epocale l'aver introdotto il principio del silenzio-assenso nel caso in cui la Regione competente si astenga dall'emettere il proprio parere entro dodici mesi dalla trasmissione da parte dell'ente parco; venticinque anni soltanto otto parchi nazionali hanno ottenuto l'approvazione dei piani da parte delle Regioni competenti. ogni legge è perfettibile, e l'ottimo forse è nemico del buono. Noi riteniamo che questo provvedimento sia comunque migliorativo del contesto generale e, quindi, lo sosteniamo.

finalmente la modifica della legge n. 394 del 1991, storico riferimento legislativo sulle aree protette, con l'approvazione oggi da parte dell'Assemblea del Senato, raggiunge un traguardo importante nel suo *iter* parlamentare. Devo sottolineare come questa legislatura stia rivolgendo un'attenzione molto importante alle tematiche dell'ambiente e alla sua tutela. Voglio ricordare anche l'approvazione, pochi mesi fa, del collegato ambientale.

del rapporto con la natura da parte della popolazione mondiale. Oggi si parla di *green economy* e di tutela della salute sempre più legata alla tutela dell'ambiente in cui viviamo. Le aree protette quindi poter essere inserite di diritto in questa nuova concezione di integrazione positiva del ciclo della vita dell'uomo e di tutti gli esseri viventi con la natura che ci accoglie e ci circonda. considerare è la presa d'atto, finalmente, che tutte le aree protette non possono essere poste sotto una campana di vetro, avulse da tutto l'ambiente che le circonda e, soprattutto, dall'attività dell'uomo. molto spesso proprio l'attività umana, ad esempio quella agropastorale, ha permesso, con un'armonica e rispettosa presenza nei nostri meravigliosi territori, una vera e propria tutela della flora e della fauna e lo sviluppo nei secoli di

con la necessità di tutelare l'ambiente. Si tratta di una forma di gestione più moderna e intelligente, al fine di consegnare alle generazioni future una natura sempre più protetta e di promuovere un'educazione alla sostenibilità e alla valorizzazione dei territori e delle economie locali.

sottolineare un paio di aspetti concernenti le autonomie alpine. Il provvedimento in esame riconosce importanti aspetti.

si andrà a ridurre non solo la distanza fisica, ma anche la lontananza che, in alcuni casi nel corso degli anni, è stata caratterizzata da rapporti tesi tra le popolazioni locali e l'ente parco. In prospettiva, lo spostamento delle sedi potrà anche rappresentare un'occasione occupazionale per quei giovani eroici e le loro famiglie che vivono nelle nostre aspre vallate del Piemonte e della Valle d'Aosta, continuando a credere nella sopravvivenza della nostra civiltà alpina.

Concludo con un ringraziamento particolarmente sentito per il lavoro svolto, principalmente al relatore, senatore Massimo Caleo,

e al consigliere De Salvo, con tutta la struttura della Commissione. Permettetemi, non ultimo, di fare un ringraziamento particolare al sottosegretario Barbara Degani,

Presidente, anche oggi nelle dichiarazioni di voto molti hanno richiamato l'importanza dell'approvazione, venticinque anni fa, della legge sulle aree protette;

convinzione: abbiamo avuto moltissimi casi in cui amministrazioni e Comuni che erano esclusi dal perimetro del parco chiedevano di entrarvi. Infatti, come ho sostenuto varie volte, il sistema dei parchi ha rappresentato per il nostro Paese un motore

uno strumento preziosissimo. I parchi hanno impedito la distruzione dei paesaggi più pregiati, hanno svolto il ruolo di custodi di un patrimonio di risorse ambientali che è insostituibile e che è la nostra possibilità di vita.

Ho sperato che, nel lavoro d'Aula, la questione fosse affrontata e risolta veramente. Abbiamo ottenuto piccoli risultati, nel senso che il fondo è stata diviso in

e non possiamo assolutamente accettarlo, perché riguarda proprio l'impostazione con cui ci si è voluti approcciare all'intervento sulla

da interessi locali. Doveva essere rafforzata l'impostazione che vedeva una rappresentanza degli interessi generali e diffusi, delle competenze e dell'impostazione scientifica. Competenze, interessi generali

che veramente balza agli occhi è che si è fatta un'operazione completamente all'inverso; per cui la *governance* dei parchi, ahimè, è stata messa al servizio

avesse indicato, nella *governance* degli enti gestori, direttamente i Comuni, non avremmo avuto in questi venticinque anni i risultati che sappiamo. Dobbiamo riconoscerlo: le conflittualità che ci siamo trovati di fronte in questi anni sono state esattamente quelle che vedevano, purtroppo, contrapposte un'idea un'idea magari sbagliata di sviluppo (che proveniva da amministrazioni comunali) e il parco stesso. Il parco ha rappresentato invece la possibilità di conservare, tutelare e mettere in campo idee di sviluppo completamente diverse e produttive

i parchi avevano bisogno di altro, ovvero di risorse, di strutture, di competenze e di investire in una *governance* all'altezza dei tempi che viviamo.

Petris si dovrà rassegnare: ritengo che entro il 2016, con il Governo Renzi-Alfano, avremo una nuova legge, che peraltro è una buona legge, che regolerà il sistema per i prossimi anni.

25 audizioni, 36 sedute, innumerevoli convegni, che qui a Roma e su tutto il territorio nazionale hanno alimentato un dibattito, non solo nella politica e tra la politica, ma tra la politica, le organizzazioni ambientaliste e anche gli enti gestori dei parchi e le comunità locali,

Certo, questo lungo *iter* ci dà idea della complessità della norma e dei temi che si affrontano con la stessa. Sicuramente poteva venire fuori anche un testo migliore.

Chi immagina che il mondo sia come lo si desidera può prendere delle grandi tranvate, come qualche giornale tranvate, come qualche giornale di fama internazionale nell'ultima vicenda elettorale americana, dove tutti gli opinionisti immaginavano un mondo a propria somiglianza, salvo poi scontrarsi con la realtà. La realtà è, infatti, ben diversa e l'*iter* legislativo lo sta a dimostrare: si confrontano tesi diversi; vengono fuori argomentazioni diverse e alla fine si arriva alla composizione delle norme

siamo arrivati a questo risultato non solo dal punto di vista normativo perché, nel prospettare le potenzialità del parco e dell'ente parco in genere,

Abbiamo ridefinito in maniera positiva il ruolo del presidente del parco, che a mio avviso viene significativamente rafforzato. Abbiamo dato trasparenza alla questione questione della nomina dei direttori dei parchi, che erano diventati una sorta di casta e di *lobby* chiusa. Invece, abbiamo fatto in modo che possano emergere in maniera positiva nuove figure e nuove professionalità. Abbiamo esaltato il ruolo del comitato tecnico nazionale e abbiamo definito esattamente il significato del piano del parco con quanto ne deriva.

e unicità in tutta Europa. Credo che sia il delta più grande che esista in Europa. Sicuramente lì ci sarà un intervento importante delle comunità locali e ci sarà un ruolo di codecisione fondamentale delle Regioni.

cosa (mi dispiace che la collega De Petris sia andata via): non è mai buona politica né positivo atteggiamento avere certezze così assolute. Chi nella vita ha certezze assolute, evidentemente è portato tremendamente al rischio dell'errore e questo rischio diventa molto spesso una certezza. Mi rendo conto che nelle letture giovanili della collega De Petris e di altri colleghi che sono alimentati da questo sacro fuoco delle certezze non ci siano stati gli scritti di sant'Agostino,

le esigenze di interessi che molto spesso appaiono confliggenti. A questo proposito, vorrei concludere esprimendo un mio parere personale che probabilmente non impegna neanche tutto il Gruppo al quale appartengo: dobbiamo finirla di immaginare in maniera demoniaca la figura di quanti esercitano l'attività venatoria. Chi esercita l'attività venatoria, infatti, è nella quasi totalità

È quindi di tutta evidenza il fatto che dobbiamo interpretare la figura di chi esercita l'attività venatoria come un tutore dell'ambiente, anche perché - diciamolo con molta franchezza se così non fosse, entrerebbe in una confliggenza di interessi che poi alla fine diventerebbe autodistruttiva per l'esercizio della propria attività sportiva.

forse ci si è accorti che era una norma incostituzionale, o forse è stata introdotta proprio per poterla poi eliminare e far vedere quanto si era disponibili. accolto un ordine del giorno per conservare la competenza del Corpo forestale dello Stato presso i parchi in termini di tutela, ma l'emendamento da cui traeva origine non è stato approvato (e sappiamo quanto peso hanno gli ordini del giorno per questo Governo).

nulla di nuovo sulla *governance*, quindi l'unica certezza è che non si è voluto riflettere e ragionare su questo per quanto le opposizioni ne abbiano fatto rilievo, quindi sulle competenze nel settore della conservazione e sulla tutela della biodiversità: certezze che non si sono volute smuovere. Nulla sulla parte che riguarda l'autofinanziamento dei parchi da effettuarsi con le *royalty*, con la caccia e con la vendita del marchio,

volendo mantenere in piedi queste entrate, che il fondo fosse tutto ministeriale e vincolato a delle specifiche competenze per togliere, come già ho detto in precedenza, dall'imbarazzo gli enti gestori del parco. Perché qui c'è un evidente conflitto di interessi: mi riferisco all'interesse ad autofinanziarsi, a sostenersi, con il dare o non dare ampliamenti ad autorizzazioni o cedere il proprio marchio a chi forse non ne ha proprio i meriti. Nulla di nuovo sui silenzi-assensi; le autorizzazioni ambientali sono state scippate alla Soprintendenza. Ci assicura il relatore che su questo punto hanno sentito il Mibact e che sono tutti felici e d'accordo.

di legge perfettamente in linea con la politica del Governo (perché è dal Governo che è stato dettato), benché si tratti di un disegno di legge parlamentare che ha messo insieme più proposte che davvero, in un primo momento, hanno visto una buona discussione e la partecipazione di tutti. Ma poi, dopo essersi arenato per lungo tempo, ha preso la rincorsa con un numero imprecisato ma lunghissimo di emendamenti del relatore - dettati dal Governo secondo il mio giudizio e di subemendamenti, perlopiù tutti bocciati. Quindi i tanti emendamenti che sono stati ricordati, la grande fatica che si è fatta in Commissione è stata tutta formale. Si sono quindi inseguiti lungamente questi emendamenti del relatore, che hanno completamente stravolto la logica del lavoro di revisione che si stava svolgendo nel gruppo di lavoro della Commissione. Ci restano «le mani della politica sui parchi, sempre più ostaggio di spartizioni e interessi locali, con un presidente e un direttore che possono non sapere niente di ambiente e che si trovano esposti alle pressioni dei privati che pagano *royalty* per inquinare, costretti poi - al momento del rinnovo delle concessioni - a scegliere tra la conservazione della natura senza compromessi e la possibilità di intascare qualche euro per far fronte alle croniche ristrettezze economiche». Questo è un pezzo tratto da un commento fatto da una delle maggiori associazioni ambientaliste: quelle con cui il relatore dice di avere concertato le modifiche della legge quadro sui parchi? Mi sembrerebbe alquanto strano. Per questo e per altro ancora dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

a terra e 28.000 chilometri a mare: una dimensione tale che sicuramente crea un interesse importante per la nostra Nazione.

Superare i limiti della legislazione vigente ed oltrepassare quella contrapposizione tra la difesa dell'ambiente e lo sviluppo dell'economia dei territori: questo è il principio base che ispira la nuova legge. Va soprattutto introdotta una nuova filosofia nell'affrontare i temi ambientali per la protezione di aree che non sono solo ambientali. Una nuova concezione per le aree protette, di quale sia la loro reale funzione sul territorio e, in particolare, sull'economia e sullo sviluppo socioeconomico, soprattutto per la parte occupazionale, che essa potrà dare in tutto il Paese. Si è voluta rafforzare l'azione di sviluppo dell'area naturale protetta, garantendo la tutela delle biodiversità, del paesaggio, della flora e della fauna, armonizzandosi con lo sviluppo socioeconomico attraverso azioni di semplificazione normativa nelle attività delle aree stesse. Sono state superate le difficoltà del passato, per esempio, quelle di taluni parchi nel sostenere il territorio con i suoi prodotti, la ricettività turistica, con la conseguente assenza di azioni utili al mantenimento dell'attività umana nei territori di competenza. È stato fondamentale quindi trovare un equilibrato livello di mediazione tra due concezioni sinora contrapposte: il protezionismo ambientale e i tentativi di speculazione. Un equilibrio che con questa legge mi pare si sia trovato e che comunque vede coinvolti in maniera importante gli attori delle realtà locali. è trovata una maggiore collaborazione tra gli enti locali e le realtà ambientaliste; legge che peraltro si propone di fermare una cieca contrapposizione, che in alcuni casi è servita a mantenere solo posizioni di potere e non a realizzare gli interessi propri dei territori. Vorremmo, quindi, che questa filosofia dell'utilizzo delle zone ambientali preziose da parte dell'uomo in senso positivo continuasse e che, dopo un periodo di conflittualità (ripeto, tra estremismi della protezione ambientale ed estremismi della speculazione), ritornasse ad essere una saggia e precisa via di sviluppo economico. Superate le contrapposizioni serve quella saggezza che è presente nella legge e che ha coinvolto tutte le esperienze, le sensibilità e le partecipazioni del territorio. Ecco perché è fondamentale ora coinvolgere tutte quelle competenze e professionalità che contribuiscano alla promozione delle attività dei parchi, anche esperienze esterne al perimetro della pubblica amministrazione e di una gestione, in taluni casi, sinora troppo burocratizzata. La nuova *governance* degli enti del parco viene allargata potremmo dire agli *stakeholder* presenti nei territori. Innanzitutto gli agricoltori, che sono poi i primi custodi dell'ambiente, perché non può e non deve esistere una contrapposizione tra l'attività agricola e l'ambiente, ma deve esserci una integrazione profonda tra queste realtà. Quindi gli allevatori, tante manifestazioni hanno fatto in Sardegna contro il parco del Gennargentu per una fruizione efficiente del territorio; fruizione ed anche controllo del territorio, perché allevatori e agricoltori hanno sicuramente anche una funzione importante nel controllo del territorio, non ultimo per il problema degli incendi che tutti quanti noi in Sardegna conosciamo. Indubitabile quindi l'importanza della conservazione dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico da parte di chi si dedica alla coltivazione della terra. terra. Su questi temi si sono giocate le sfide delle competenze che sono state messe a disposizione della guida dei parchi con attenzione all'interesse dell'ambiente.

Veramente grande è la rilevanza delle aree protette sull'ambiente del nostro Paese e bisognerà incentivare sia il ripopolamento delle specie animali, che quello dell'uomo. Con questo non intendiamo che vengano portate avanti speculazioni di alcun tipo, ma promossi il recupero e l'utilizzo responsabile, ad esempio, di vecchi fabbricati rurali per attività turistiche, che vadano a integrarsi nella economia delle aree dei parchi. Quello che ci preme sottolineare è che con questo disegno di legge finalmente vengono meno le diffidenze tra enti locali ed enti parco e riprende un dialogo tra chi si occupa del governo del territorio e chi di quello dell'ambiente. La *governance* dei parchi viene snellita, cessano i commissariamenti e le mancate intese. Diventa più forte la figura del Presidente del parco, che prevede l'intesa della Regione in cui insiste il parco stesso. Tale figura viene identificata da una terna di comprovata esperienza e qualificazione diventa incompatibile con le cariche elettive e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici. Stessa cura verrà posta in essere per la in essere per la composizione del consiglio direttivo, composto da sei a otto membri, che sarà designato per il 50 per cento dalla comunità del parco e avrà il compito di nominare il direttore del parco stesso. Non si perderà, quindi, il contatto con il territorio. Certo, dispiace che non siano stati accolti diversi emendamenti, tendenti a migliorare la legge in esame. Questo non vuole dire che l'obiettivo di migliorare la legge n. 394 non sia stato perseguito e pertanto, a nome del Gruppo di Forza Italia, annuncio il voto favorevole. Egregio Presidente, gentile Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo arrivati, al termine di un percorso lungo e partecipato, a discutere finalmente in Aula le modiche alla legge n. 394 del 1991. Di questo risultato voglio ringraziare, oltre al Ministro, alla sottosegretario Degani Degani e a tutti i componenti la 13a Commissione (a partire dal presidente Marinello), innanzi tutto il relatore, il collega Massimo Caleo, che con passione, competenza e tenacia ha portato avanti dall'inizio alla fine questo grande lavoro. È un altro tassello delle riforme che va al suo posto, perché, che lo si voglia o no riconoscere, il Parlamento che ha legiferato di più in materia ambientale, portando a termine ciò che nelle scorse legislature non era stato possibile fare, è proprio questo. Si è parlato tanto nei giorni scorsi di questa riforma, anche a sproposito, con l'obiettivo di distorcere la realtà delle cose e opporsi al cambiamento di una legge strategica come la n. 394, che aveva, certo, dato buona prova di sé in questi venticinque anni, ma che senza dubbio doveva essere aggiornata e corretta per corrispondere al meglio al fine ultimo per il quale era stata approvata: cioè, regole chiare per tutelare fauna e flora in aree di pregio ambientale e farle diventare un'opportunità di sviluppo di quei territori nella legalità. Sì, nella legalità, perché ce lo hanno chiesto in tanti Presidenti di parchi nazionali; presidenti come Giuseppe Antoci, che in quel ruolo sta rischiando personalmente la vita svolgendo un presidio importante di legalità e che saluto con calore, perché è presente ai nostri lavori. Dall'ottobre 2014, quando è stato incardinato il testo unificato in Commissione, si è svolta una discussione ampia e articolata, preceduta dall'ascolto di decine di portatori di interesse, senza alcuna esclusione, a cui è seguita la fase propositiva da parte dei colleghi con migliaia di emendamenti presentati, discussi e molti dei quali accolti. Il testo unificato, quindi, giunge in Aula modificato in modo importante da un confronto, una mediazione e una condivisione tra le diverse forze politiche, che qui in Aula, ancora una volta, si preoccupano più di tutto di differenziarsi e distorcere la realtà

e del Governo, che purtroppo non è stata colta, né riconosciuta dalle dichiarazioni di voto finale, spesso pregiudiziali, da parte di alcune forze politiche. Ma cosa sono oggi i parchi nel nostro Paese? Molto semplicemente si potrebbe dire luoghi di bellezza e laboratori di sviluppo che tutte le istituzioni dovrebbero valorizzare maggiormente come parte essenziale della propria identità e ricchezza. La parola «parco», infatti, pur non comparendo in alcun articolo della nostra Costituzione, trova piena corrispondenza nei valori interpretati oggi dalla loro attività e identità dentro l'articolo 9, tra i principi fondamentali, dove si sancisce che: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. il presidente Ciampi che la presenza tra i principi fondamentali di questo articolo «offre un'indicazione importante sulla "missione" della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli». Ecco quindi il senso vero di questa scelta: una missione, un modo di vivere e di pensare a cui la legge n. 394 ha dato un corpo e gambe su cui poter crescere e camminare. Ora serve farlo meglio, con strumenti più adeguati e al passo con i tempi, che non vedano più la visione altra dei parchi rispetto al contesto nel quale sono inseriti, ma sempre più integrata e in relazione con le altre istituzioni, con le imprese, la società civile e il privato sociale. trovare soluzioni più avanzate, senza timidezze o incertezze, per rafforzare la legislazione sui parchi, perché il loro futuro è legato a doppio filo con la qualità e la competitività del sistema Italia. Per questo merita risposte all'altezza, per dare il senso che anche questo ambito strategico può e deve essere una risposta innovativa alla crisi economica che stiamo vivendo. Di queste risposte all'altezza della sfida, la legge che approveremo oggi ne contiene tante. Ne voglio ricordare solo alcune tra le più significative. luogo, si è messo mano alla *governance* dei parchi per superare anacronistici metodi di nomina dei Presidenti, che non avevano prodotto il risultato voluto ma spesso stalli e commissariamenti prolungati, con metodi che nulla sacrificano sulle competenze, allargando invece a figure in grado di mettere a disposizione professionalità gestionali di enti complessi, che sono sempre più necessarie. Si è intervenuti per superare l'albo dei direttori, in coerenza alla riforma della pubblica amministrazione che ha introdotto il ruolo unico per i dirigenti pubblici, aprendosi a nuove competenze finora escluse e generabili solo con la selezione pubblica. allargata la rappresentanza nei consigli ai portatori di interesse delle comunità dei parchi, a partire dai sindaci, - sì, i sindaci, che continuano ad essere la massima espressione diretta dei cittadini - e coinvolgendo il mondo dell'agricoltura che in questi ultimi vent'anni è stato il più valido alleato dei parchi, permettendo di coniugare la tutela dell'ambiente con l'agricoltura di qualità e le produzioni tipiche certificate, la legalità e l'economia di filiera. Come si vede e si può leggere nel testo, non c'è alcuna deriva localistica né una dequalificazione delle competenze, ma solo una scelta - per dirla con un termine non più nuovo - *glocal*: una una valorizzazione delle comunità locali, per rendere più forte e incisivo il pensiero globale sui parchi. In secondo luogo, ci siamo preoccupati di migliorare gli strumenti e le misure per la tutela della biodiversità a questo da parte della collega De Petris, anziché perdersi in dissertazioni campate per aria sul dopolavoro di qualcuno. Vengono affidate alle pianificazioni ambientali degli enti di gestione dei parchi anche le aree della rete Natura 2000, i siti di interesse che siano ricomprese o anche solo contigue al territorio del parco senza modificare le norme di tutela e prevenzione, prevedendo l'estensione a mare dei parchi terrestri confinanti con aree marine protette per chiarire e definire in modo omogeneo le azioni di tutela da perseguire, includendo le aree contigue nella pianificazione del parco con le Regioni (e non più su iniziativa di queste ultime, cosa che aveva creato una situazione assolutamente disomogenea nel Paese), riscrivendo le modalità di gestione della fauna selvatica, che sanciscono una volta per tutte e per le legge il divieto di caccia nelle aree parco, e prevedendo una gerarchia nelle modalità di intervento per l'eradicazione delle specie dannose e alloctone. Una gerarchia che passerà prima dai metodi non cruenti, laddove possibile (metodi che con questa legge vengono finanziati per la prima volta in modo permanente), per arrivare alla caccia di selezione con personale adeguatamente formato, previo parere vincolante dell'ISPRA (non sulle aree contigue, dove non c'era mai stato)

La terza questione riguarda le risorse e i beni dei parchi. Per la prima volta, dopo l'approvazione della legge n. 221 del 2015, meglio nota come collegato ambiente, diamo attuazione alla previsione sulla valorizzazione economica del capitale naturale, dei cosiddetti servizi ecosistemici. Lo facciamo in due modi: introducendo, da un lato, una delega al Governo per individuare criteri e metodi univoci per remunerare i diversi servizi e, dall'altro, prevedendo *royalty* per la prima fase di applicazione. Saranno risorse destinate ai parchi, sia nazionali che regionali, al 50 per cento, da prelevare ai titolari di reti energetiche

ci siamo preoccupati di trovare una soluzione per i beni demaniali inutilizzati. Da ultima, ma non per importanza, la scelta fatta sulla semplificazione burocratica. Nella mia passata esperienza di presidente di un parco regionale dell'Emilia-Romagna - mi rivolgo alla collega De Petris, che ha parlato di dopolavoro di qualcuno: a differenza di lei, qualcuno in Commissione una esperienza passata nel merito l'aveva fatta - al primo posto nelle lamentele dei cittadini e delle imprese residenti ci sono sempre state le lungaggini amministrative nel momento in cui vi era la necessità di mettere mano all'edificato esistente. E noi cosa facevamo, di fronte al cittadino o all'impresa? Ci presentavamo con tre soggetti diversi (il comune, l'ente parco e la soprintendenza). Oggi si passerà ad una pianificazione condivisa del parco con la soprintendenza e con la Regione, dopo la quale sarà l'ente parco stesso l'unico soggetto titolato a rilasciare il nulla osta paesaggistico. Si tratta di una vera rivoluzione per chi ha vissuto, anche solo indirettamente, i ritardi della situazione attuale. Non sarà la risoluzione di ogni problema, ma è una soluzione innovativa, per coniugare assieme le esigenze di tutela con quelle di efficacia dell'azione amministrativa e di valorizzazione dei beni. Consegniamo, quindi, un buon lavoro alla Camera dei deputati, frutto di un confronto ampio, che ci auguriamo non venga stravolto e, se ci saranno le condizioni, possa diventare legge quanto prima. È una buona revisione della legge n. 394 con la quale possiamo riposizionare il nostro Paese a livello storia, tutela, biodiversità, semplificazione, innovazione e sviluppo sono le parole chiave di questa scelta. Ne aggiungo solo una: la lungimiranza. Significa non gestire l'esistente, ma provare ad anticipare il futuro. Come fece nel lontano 1980 un amministratore locale del mio territorio, il professor Liliano Famigli, che ci ha lasciato troppo presto pur insegnandoci tanto, quando decise, assieme a tecnici preparati come lui, di istituire l'assessorato provinciale all'ambiente, sei anni prima della costituzione del Ministero dell'ambiente. Fu una scelta che consentì di sviluppare importanti programmi, spesso pionieristici. Liliano scriveva: «Una nuova concezione della politica ambientale è quella che non separa l'uomo dalla natura, e da questo dipenderà in larga misura, non solo la futura qualità della vita dei nostri territori, ma anche la possibilità di assicurare la crescita produttiva È con l'ambizione di essere lungimiranti come lo fu lui e tanti altri amministratori del nostro Paese che annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

come possiamo vedere, gli ordini del giorno che danno un piccolo contentino, per poter immaginare che qualcosa si faccia. Ma qual è il vero problema di questa

Comunico che è stata sottoposta alla Presidenza, dal richiesto numero di senatori, una proposta di inversione dell'ordine del giorno

Abruzzo. Il Parlamento ha provato a raccogliere le proposte venute da diversi Gruppi politici, unificandole nel presente disegno di legge, per dare vita ad una Commissione d'inchiesta sulla risposta all'emergenza e il processo di ricostruzione che è tutt'ora in atto. Ci lasciamo alle spalle, come i colleghi sanno, anni duri per gli abruzzesi e per le istituzioni che li rappresentano, che hanno dovuto fare i conti con una serie di problematiche, con difficoltà rispetto alla *governance* così come si è evoluta nel corso del tempo e con l'assenza di regole certe nell'immediato e risorse costanti. Si è dovuto attendere parecchio tempo prima di conoscere quelle che poi sono state indicate come le linee guida e le procedure per la ricostruzione delle case danneggiate dal sisma. Si tratta di lentezze e ritardi che hanno costretto la ricostruzione a stentare nell'avvio

all'infiltrazione di organizzazioni criminali nel processo di ricostruzione, come testimoniano le diverse inchieste giudiziarie aperte nel corso di questi anni e i vari moniti sollevati anche di recente dal procuratore distrettuale antimafia dell'Aquila, Fausto Cardella.

dei diversi atti, da quello a prima firma della senatrice Stefania Pezzopane a quello a prima firma del senatore Maurizio Romani, a quello presentato dalla senatrice Blundo, scegliendo come più utile e e più immediata la forma della Commissione monocamerale, cui vogliamo affidare compiti di indagine, oltre a condividere la maggior parte di quelli proposti dai disegni di legge iniziali, che abbiamo integrato a chiarito durante la discussione in Commissione.

sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sull'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie e sul termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione, sul complesso delle risorse stanziate, alla data del 31 dicembre 2015, che fanno riferimento ad altri sismi

dell'emergenza, la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali. Ci sono poi altri punti, l'ultimo dei quali è stato aggiunto in Commissione su richiesta

un insieme di previsioni, compiti e funzioni che vengono affidati a questa Commissione che dovrà essere formata da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato proporzionalmente al numero di componenti di ogni Gruppo parlamentare e comunque assicurando La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a tutti i procedimenti e le inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti

limitandomi ad aggiungere alcune considerazioni. Il testo che è stato approvato in Commissione è assolutamente agile e snello e comprende, a mio avviso, diversi aspetti delle questioni legate alle grandi calamità del nostro Paese e, in particolare, alla calamità che ha colpito gravemente L'Aquila e altri 56 Comuni nel 2009.

(tra l'altro allora erano bicamerali) sul terremoto del Belice e non si è mai arrivati a una conclusione; anzi, peggio, le conclusioni dell'ultima Commissione del 2001 non sono servite minimamente a supportare alcuna iniziativa parlamentare o governativa che potesse mettere la parola fine a questa antica questione. Il nostro auspicio oggi, invece, è che lo strumento versatile della Commissione monocamerale possa produrre un buon lavoro, che, a mio avviso, non deve guardare prevalentemente all'aspetto delle colpe o della responsabilità. Quelle sono competenze che spettano ad altre istituzioni o ad altri organismi. Sono convinto che oggi il compito principale sia quello di fotografare lo stato dell'arte e soprattutto trovare soluzioni, nei tempi e nei modi che si vorrà individuare, per dare una risposta compiuta a quelle popolazioni, al fine di dare un segnale importante per l'intero Paese, specie in un momento come questo in cui purtroppo il dramma del terremoto continua a fare vittime, a produrre guasti e a flagellare gran parte del territorio nazionale.

rinuncerò a intervenire in fase di dichiarazione di voto, perché credo di aver esaurito gli argomenti in questo unico intervento.

È importante fare chiarezza, non solo per le ingenti quantità di risorse dell'erario pubblico spese, ma soprattutto per dare

dovrà occupare anche degli eventi che hanno riguardato la ricostruzione successiva ai sismi «nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012,

al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate» lo sottolineo in maniera molto particolare «dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche».

che ha colpito la Valnerina, interventi fatti dopo il 1997, che in alcuni casi non hanno prodotto gli effetti di resistenza che ci si sarebbe aspettati. Occorre fare chiarezza, per capire ciò che è stato, ma soprattutto per costruire un percorso, un protocollo, una modalità operativa che rendano efficaci le risorse spese

verificate tutte le modalità con cui impedire, fino al limite massimo che sia possibile immaginare, che questi eventi possano essere infiltrati. Si tratta di un compito impegnativo e su questo valuteremo il lavoro della Commissione. In via preliminare non possiamo che essere favorevoli a che si faccia chiarezza e, anzi, auspichiamo che la si faccia in termine

delle decisioni politiche del Senato stesso e non viceversa. Pertanto, se ci sono delle questioni di spesa devono essere subordinate alle questioni istituzionali. Questo andrebbe fatto sempre: non solo quando si parla di questa Commissione d'inchiesta - lo dico con una piccola vena polemica - ma anche quando si tratta di riforme costituzionali.

coperte dai risparmi che continuano ad essere effettuati anno per anno, sommando risparmio a risparmio. Dal punto di vista degli spazi, essi saranno, per forza di cose, limitati, non sarà facile trovare la migliore delle sistemazioni, ma sono convinto che lo spirito di servizio e l'interesse per il contenuto di questa Commissione d'inchiesta saranno prevalenti.

trovare tutte le soluzioni utili allo svolgimento di queste funzioni nel limite delle disponibilità di risorse e di spazi del Senato. PRESIDENTE. Ha facoltà Signor Presidente, onorevoli senatori, l'approvazione dell'istituzione della Commissione d'inchiesta monocamerale sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 è un passo importante per ristabilire la reale portata di quanto accaduto a seguito del terremoto aquilano, per evitare in futuro lentezze, inefficienze e ritardi. Lasciatemi dire che l'istituzione di questa Commissione deve essere l'occasione per analizzare quanto successo ma soprattutto per capire, approfondire ed evidenziare - come ha detto bene il senatore Marinello - quali possono essere le procedure più corrette da porre in essere in casi di disastri naturali che cominciano, ahinoi, ad essere sempre più frequenti nel nostro Paese: non è pensabile che possano trascorrere sette anni, come quelli vissuti in Abruzzo, con l'assenza di regole certe per la gestione dell'immediato e in attesa di linee guida e di ordinanze che consentano di destinare correttamente e celermente le risorse messe a disposizione. La strada maestra, anche alla luce degli ultimi avvenimenti tellurici che hanno colpito il Centro Italia, deve essere quella di porre in essere prima azioni e provvedimenti che mirino a salvaguardare la nostra gente e il nostro territorio e a intervenire celermente nelle situazioni emergenziali e *post* emergenziali delle grandi calamità naturali. La relazione della 13a Commissione - come ha detto bene il senatore Vaccari - va nella giusta direzione quando osserva che le modalità di intervento per la ricostruzione *post* sismica devono prendere una nuova strada di garantismo e di velocità, evidenziando come l'attesa delle linee guida e il susseguirsi di ordinanze abbia di fatto rallentato il processo di ricostruzione ricostruzione che ancora oggi non è del tutto terminato. Per tutti questi motivi ribadiamo come l'istituzione di una Commissione possa rappresentare l'opportunità di capire e di entrare nel cuore del problema, sviscerando una metodologia chiara che ci aiuti ad affrontare la ricostruzione. Se non riusciremo a fare ciò, potremo istituire altre Commissioni di inchiesta che non faranno altro che accertare le nuove responsabilità, ma la loro istituzione sarà solo la manifesta prova - come è stato detto da molti autorevoli senatori - dell'incapacità di risolvere i problemi nel momento in cui si verificano.

indagare anche sull'adeguatezza della pianificazione strategica adottata dal Comune. Noi, allo stato attuale, vediamo che il centro storico dell'Aquila non è in condizioni di essere utilizzato, tant'è che con le ultime scosse è stato nuovamente chiuso. Vediamo che ci sono delle ricostruzioni di edifici che hanno priorità rispetto ad altre e non c'è chiarezza su questa priorità per la possibilità di ripresa dell'intera città e, soprattutto, del suo tessuto economico. Quindi una valutazione sull'adeguatezza di questa pianificazione strategica è forse necessaria, soprattutto perché per i nuovi centri storici colpiti dai terremoti degli ultimi giorni si devono valutare quali sono i giusti interventi e le giuste priorità da assegnare per la ricostruzione.

ritengo opportuno perlomeno tentare di invitare quest'Assemblea a considerare in modo diverso questi emendamenti. In questo caso parliamo di un sito di stoccaggio che è stato considerato come unico

le prime ore di ciò che è accaduto e con delle modalità molto particolari. Era intervenuto anche l'Esercito per ripristinare quel sito che versava in condizioni non idonee.

ha colpito duramente l'Abruzzo con una magnitudo di 6,3 della scala Richter, con un epicentro a poco più di un chilometro dal centro dell'Aquila. Il bilancio fu drammatico: 309 vittime, migliaia di feriti, distruzione del centro storico e di interi quartieri della città, capoluogo della Regione Abruzzo, e di 57 paesi della Provincia, il cratere, con migliaia di sfollati. Ricordo bene come simbolo e memoria di quel sisma furono quei 55 ragazzi studenti morti, ospitati nella casa dello studente, dove una parte della palazzina crollò sbriciolandosi. Quello dell'Aquila è uno dei tanti eventi di calamità naturale che nel corso della storia, anche recentissima, hanno colpito il nostro Paese. Purtroppo, però, anche in questo *post* terremoto si sono manifestate opacità e malagestione delle risorse. Voglio qui ricordare ai colleghi dell'Aula del Senato che sono stati già spesi 11 miliardi e che altri 7 se ne aggiungeranno.

che si sono costituiti anche in associazione, è doverosa dunque la trasparenza ed è doveroso creare le condizioni per garantire giustizia. A sette anni e mezzo dal sisma, la ricostruzione è ancora in atto. Pensate che l'altro giorno con toni entusiastici diciamo francamente infelici - all'Aquila è stata fatta l'inaugurazione del primo cantiere in 13 frazioni, mentre nelle altre 30 frazioni è ancora in alto mare e se va bene, nella seconda metà del 2018 partiranno i primi cantieri. Senza contare il problema dei sottoservizi, dove non ci sono certezze, non ci sono fondi e non ci sono progetti. Infatti, i cittadini e le istituzioni lamentano ritardi, lentezze ed inefficienze. L'ultima novità è proprio dell'altro giorno all'Aquila, dove per un avviso pubblico, mal comunicato dall'amministrazione comunale, oltre 720 famiglie che hanno fatto richiesta per essere rimborsati dai danni provocati da quel terremoto sette anni e mezzo fa ai loro mobili, probabilmente non riceveranno mai questi soldi. La confusione e la contraddittorietà delle norme emanate spesso hanno dato luogo ad azioni della magistratura amministrativa, penale e contabile che, in particolare, hanno visto ricadere la responsabilità sugli amministratori locali impegnati nella ricostruzione. Le inchieste della magistratura evidenziano episodi di corruzione e tentativi di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel processo di ricostruzione che, ovviamente, ha attirato elevati interessi economici, legali e illegali. La Commissione d'inchiesta parlamentare monocamerale dovrà, dunque, occuparsi delle problematiche connesse al periodo di emergenza e anche alla ricostruzione. Il nostro Gruppo ha contribuito convintamente al miglioramento del testo.

(non, dunque, solo alla fase dell'emergenza, che era la prima ipotesi); la possibilità di indagare sulle misure di sicurezza adottate nelle aree colpite dal sisma, allo scopo di verificare i reati commessi contro il patrimonio immobiliare abbandonato, pubblico e privato, e a danno delle persone; la possibilità di indagare sulle misure adottate nell'ambito della ricostruzione, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza antisismica degli edifici e della tutela ambientale; la verifica dello stato in cui versano oggi gli immobili del progetto CASE per la scarsa o assoluta mancanza di manutenzione; l'ampliamento delle indagini sulle responsabilità nei collaudi effettuati nelle diverse fasi di costruzione; l'ampliamento delle attività della Commissione d'inchiesta, comprendendo anche indagini sulla gestione delle risorse stanziate con provvedimenti successivi a quelli dell'emergenza (quindi anche i successivi decreti-legge). nostra proposta, accettata, è la possibilità per la Commissione di svolgere indagini sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisionali realizzate nei centri storici, come, ad esempio, i puntellamenti degli immobili dissestati. Con questa Commissione d'inchiesta il Parlamento, il Senato - essendo la Commissione monocamerale - ha una grande responsabilità nell'individuare le problematiche connesse alla ricostruzione e per portare alla luce le patologie emerse sia nell'emergenza sia, soprattutto, durante la ricostruzione. Ci auguriamo che le indagini svolte dalla Commissione possano contribuire non solo alla correzione delle misure fin qui adottate per la ricostruzione del territorio dell'Aquila e dei Comuni del cratere, ma anche al perfezionamento di un modello di intervento che si è già voluto con il terremoto di Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto del 24 agosto scorso e che, come Curcio (il capo del Dipartimento della protezione civile) ha detto in audizione l'altra sera, già necessita di una rivisitazione a seguito delle scosse del 26 ottobre e di quelle del 30 ottobre, con magnitudo 6,5. Questo ovviamente per far fronte in futuro - si auspica - con maggiore efficienza ed efficacia alle fasi di emergenza e di ricostruzione di zone colpite da calamità naturali che, purtroppo, periodicamente colpiscono - e,

credo che, benché siano passati oltre sette anni da quella notte del 6 aprile 2009, 2009, sia comunque assolutamente necessario che il Senato possa meglio indagare. Non a caso, tra l'altro, questa proposta ha raccolto suggerimenti provenienti da diversi Gruppi politici

che la Commissione riesca a comprendere fino in fondo i ritardi, le lentezze, il sistema di *governance* che si è messo in campo nella fase di ricostruzione. Credo infatti che ciò possa aiutarci a non ricommettere gli stessi errori, che possa rendere assolutamente solerti le istituzioni nei meccanismi di controllo.

sono tenute o che sono in via di formazione in questi ultimi mesi, forse arriva un po' tardi. Infatti credo che avremmo potuto deliberare con molta più rapidità,

(situazione che mi provocò un grande dispiacere al punto da scrivere, in modo inadeguato e equivocabile, un *tweet* del quale mi scuso nuovamente), avevano provocato in me grande delusione. Oggi, finalmente, alla luce anche dei nuovi pericoli e del nuove sciame sismico che sta colpendo l'Italia centrale, esprimo la mia più viva soddisfazione per l'accoglimento da parte di tutti i Gruppi della richiesta, avanzata dal mio Gruppo, di inversione del calendario, permettendo di fatto il completamento oggi in Aula dell'*iter* relativo alla costituzione della Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione *post* sisma della città dell'Aquila. È questo un passo importante, fortemente voluto dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle che da sempre ha appoggiato la mia proposta di istituzione di questa Commissione. Si tratta - lasciatemelo dire - del raggiungimento di un importante traguardo personale, oltre che politico, che ho inseguito con tutta me stessa fin dall'inizio del mio mandato parlamentare. Un obiettivo grazie al quale si potrà finalmente fare chiarezza sulle responsabilità politiche e le motivazioni che hanno ritardato il processo di ricostruzione, attualmente ancora caratterizzato da notevoli rallentamenti nel capoluogo abruzzese, soprattutto per il centro storico della città, e la mancata ricostruzione dei centri storici del cratere, nonché sulle modalità poco trasparenti che hanno caratterizzato in questi anni la gestione delle risorse stanziate, con numerose situazioni e appalti per la messa in sicurezza e la ricostruzione che sono finti sotto la lente di ingrandimento

che indaghi sulla tipologia e la qualità dei materiali utilizzati, nonché sulle fasi di progettazione, manutenzione e collaudo degli immobili ricostruiti, contribuisce anche il fatto che molte abitazioni aquilane, appena restituite ai proprietari a sette anni e mezzo dal terremoto, hanno subìto dei nuovi danni dallo sciame sismico del 24 agosto sebbene non siano state dichiarate inagibili o pericolose per la popolazione. Ho iniziato la mia battaglia di chiarezza e trasparenza sull'utilizzo dei fondi stanziati per la ricostruzione dell'Aquila fin da quando emersero le prime anomalie, i primi appalti gonfiati, le prime ingiustizie, i primi casi di infiltrazione mafiosa e di corruzione nella gestione dei fondi: fondi per una popolazione già già perseguitata e prostrata dagli eventi drammatici del terremoto. In settantotto mesi sono stati stanziati quindici miliardi di euro, ma sul completamento dei lavori di ricostruzione molta strada deve essere ancora fatta. Quello che si è presentato agli occhi degli aquilani in questi anni, cari colleghi, è un quadro agghiacciante, un intreccio perverso di interessi che ha visto e vede coinvolti politici, funzionari, imprenditori, tutti disinvoltamente capaci di muoversi all'interno della perversa logica del *do ut des*. Uniche vittime i cittadini onesti, quelli che aspettano ancora la ricostruzione degli edifici residenziali pubblici e di alcune importanti strade dell'Aquila, come via Aldo Moro, ha subìto dei danni che l'hanno resa inutilizzabile. Molti di quelli che aspettano la rinascita della nostra amata città hanno difficoltà a vedere riconosciuti i loro diritti. L'accertamento delle responsabilità politiche nazionali e locali per lo stato di crisi in cui versa la città dell'Aquila è quindi una priorità oggi, alla luce delle numerose operazioni di polizia nonché alla luce di ciò che si deve fare per i territori colpiti e di ciò che sta accadendo all'interno delle altre realtà

provocando la chiusura di numerose attività commerciali autoctone. In questi sette anni L'Aquila è stata costretta a ingoiare molte pillole di malaffare, assistendo impotente allo sgretolamento

A San Gregorio si è addirittura provveduto allo sgombero di molte famiglie, dopo averle fatti vivere per sette anni in case lesionate e parzialmente agibili, senza provvedere, come per altro accaduto per gli edifici residenziali pubblici di via di Vincenzo, all'impiego effettivo delle risorse pubbliche stanziate appositamente per la loro ricostruzione e facendo aprire alla magistratura l'ennesima inchiesta. Si tratta di alloggi di proprietà privata e quarantanove di edilizia residenziale pubblica del comune dell'Aquila ed è stata pagata una rata di circa un milione e mezzo, senza che i lavori siano mai iniziati. L'emergenza e la disperazione dei settantamila si è trasformata, quindi, in un grande affare per le imprese mafiose, puntualmente fallite per non rispondere di nulla, mentre i cittadini ci hanno rimesso in sicurezza e salute. Il contributo che ha dato il Movimento 5 Stelle nel chiedere la discussione d'urgenza del provvedimento si è rivelato non solo determinante, ma ha permesso anche l'accoglimento degli ulteriori emendamenti che ho presentato per la verifica dei fondi stanziati per l'edilizia residenziale pubblica e delle condizioni sanitarie e lo stato di ricostruzione dell'edilizia scolastica,

individuare le responsabilità politiche locali e nazionali per tutti i ritardi e i continui episodi di mala gestione che hanno contraddistinto le attività di ricostruzione dal 2009. Tra le funzioni della Commissione d'inchiesta, oltre a quelle di verifica sulle modalità di gestione di tutte le risorse stanziate e l'adeguatezza dei piani per la ripresa delle attività produttive, c'è anche la gestione delle macerie ed i siti di stoccaggio, la messa in sicurezza, la certificazione energetica, il risparmio idrico, i reati commessi contro il patrimonio e le infiltrazioni della criminalità e l'accertamento dello stato in cui versano oggi gli immobili del progetto CASE, le cause del ritardo dell'assegnazione dei fondi e l'esame della reale efficacia di tutta la normativa che ha disciplinato la fase della ricostruzione. Questo anche al fine di poter dare adeguate indicazioni. Un ulteriore ambito d'azione riguarderà l'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti. Per questi motivi, ringraziando ancora una volta il mio Gruppo e tutte le altre forze politiche che hanno per0messo di poter raggiungere oggi questo importante traguardo, annuncio ovviamente il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Occorre infatti garantire correttezza e trasparenza delle procedure per onorare la memoria di tante, tantissime vittime ed eliminare quel disagio che tanti, tantissimi

Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi,

del buon terremotato e sapeva cosa doveva fare per assistere, aiutare, sostenere l'emergenza e, poi, impostare la ricostruzione.

come fu gestita l'emergenza e su come sono stati fatti i primi provvedimenti. Ricordo l'affastellarsi delle ordinanze, le leggi contraddittorie e l'esclusione dal potere di decisione dei Comuni e degli enti locali fino al 2012. poi, dei provvedimenti contraddittori, la cui contraddittorietà oggi emerge ancora più plateale di fronte ai nuovi eventi sismici che hanno indotto, giustamente, il Governo a emanare un decreto-legge che fa tesoro degli errori commessi a L'Aquila e li risolve positivamente. Qualcuno durante il dibattito ha citato il ritardo nella ricostruzione dei centri storici. Nessuno, però, ha ricordato che allora il Governo e il Parlamento non vollero non vollero acconsentire alla ricostruzione finanziata delle seconde case. Ancora oggi, nel cratere del terremoto aquilano del 2009, solo a seguito di provvedimenti che questo Governo e questa maggioranza hanno adottato, è possibile ricostruire le parti comuni. Pensate che questo non abbia comportato un ritardo gigantesco nella pianificazione dei Comuni, che si sono trovati ad avere aggregati in cui la prima casa a volte era soccombente, numericamente e come cubature, rispetto alla seconda casa? sede abbiamo dovuto risolvere il problema, grazie al sostegno del Partito Democratico e alla lungimiranza del Governo e di questa maggioranza, che hanno voluto riparare ad alcuni errori, in cui non voglio vedere né colpa, né dolo:

quali siano stati gli errori in tutta la filiera e quali possano essere - è urgente dirlo al Paese - gli strumenti più idonei per lo Stato (attraverso i suoi organi: la Protezione civile e il Governo), per gli enti locali e per le Regioni che nel nuovo terremoto immediatamente assumono poteri di vice commissari attraverso i presidenti. ricevono immediatamente dei poteri e, quindi, già con i nuovi decreti‑legge si risolvono positivamente alcuni dei problemi che abbiamo avuto. i punti della proposta di legge siano tutti molto chiari e giusti. Ritengo che si farà un buon lavoro, che dovrà essere serio e breve, scevro da strumentalizzazioni di ogni tipo e unicamente finalizzato a dire al Paese, che ha sostenuto tanti sacrifici per indurci finalmente a un avvio serio della ricostruzione, perché, come e e quando si completerà questa ricostruzione, per dare poi agli altri territori, anche con una legge organica, anche con Casa Italia, gli strumenti opportuni affinché quello che è accaduto da noi non accada più a nessun altro.

di Pescara e Chieti ai dirigenti scolastici per invitare gli stessi a dare massima diffusione fra studenti e docenti a un evento nella città di Pescara: oggi alle 18, al teatro Circus di Pescara, Luca Sofri (marito della neonominata a RAI 3) intervisterà il Matteo, Presidente del Consiglio, all'interno della XIV edizione del Festival delle letterature di Pescara. Badate bene che nell'invito si dice chiaramente di assistere proprio all'intervista di Renzi e non al resto degli appuntamenti culturali che si terranno oggi e nei giorni seguenti. cosa avranno in cambio gli studenti? Un riconoscimento, formalizzato in attestato, rilasciato a chi seguirà l'intervista-propaganda. La più alta istituzione scolastica della Regione, dunque, entra a gamba tesa nella campagna referendaria, mentre il suo compito dovrebbe essere quello di coordinare la formazione in maniera neutrale e senza orientamento politico e partitico. Le province di Chieti e di Pescara sono tappezzate da raffigurazioni, in tutta probabilità in violazione del codice della strada e delle norme sulla campagna elettorale. La passerella di Renzi, affiancata alla dicitura «Basta un sì», altro non è che una prova tecnica di regime. L'invito alle nostre popolazioni è di rispondere pacificamente, democraticamente e con una straordinaria partecipazione, il 4 dicembre: a queste imposizioni antidemocratiche non si può che rispondere con un gigantesco "no".